la Conferenza dei Capigruppo, appena conclusa, ha ridefinito il calendario della settimana corrente ed ha approvato il nuovo calendario dei lavori per la prossima settimana. La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 20. Sono confermati gli orari delle sedute di domani. Entro le ore 20,30 di domani si concluderà la trattazione degli emendamenti al decreto-legge sulla sicurezza. A tal fine, sono stati rimodulati i tempi a disposizione dei Gruppi,

Le dichiarazioni di voto e il voto finale sul decreto-legge in materia di sicurezza si svolgeranno a partire dalle ore 11 di martedì 24 giugno. Nella seduta antimeridiana di giovedì 19, dalle ore 9 alle ore 13, sarà discusso il decreto-legge sul trasporto aereo, fino alla sua votazione finale che avverrà alle ore 13, secondo i tempi già distribuiti. La seduta pomeridiana non avrà luogo. La prossima settimana, nel pomeriggio di martedì 24 giugno, sarà discussa la proposta d'inchiesta parlamentare sugli infortuni sul lavoro. Nel prosieguo della settimana, sarà iscritto all'ordine del giorno il decreto-legge in materia fiscale secondo i tempi ripartiti in allegato al calendario. Sempre nel corso della settimana sarà posta all'ordine del giorno la mozione n. 9 con procedimento abbreviato sulla valorizzazione della dieta mediterranea. Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno avrà luogo il *question time*.

Lei deciderà poi sull'ammissibilità degli emendamenti di cui abbiamo discusso stamani. Ma c'è un profilo di delicatezza e di galateo istituzionale che attiene alla lettera del Presidente del Consiglio il quale, dichiarandosi

*(PD)*. Signor Presidente, buona parte degli emendamenti che abbiamo presentato sono di tipo cosmetico, se così si può dire.

apprezzabile e digeribile, una serie di norme odiose che sono al centro del cosiddetto decreto sicurezza. La sostituzione, in particolare, di alcune parole desuete o che possono trarre in inganno

che riguardano l'espulsione e l'allontanamento. Come è facile notare, sia nell'articolo 235 che nell'articolo 312 si usa l'espressione «il giudice ordina l'espulsione»,

Ed allora sembrerebbe quasi che con questa disposizione di legge si sia voluto abrogare la citata legge del 1986 e inserire di nuovo la pericolosità presunta. Se così non fosse, infatti, se effettivamente il legislatore non avesse ignorato quella legge o non l'avesse voluta ritenere superata, avrebbe usato espressioni diverse. Invece che «il giudice ordina l'espulsione» avrebbe dovuto usare l'espressione «il giudice può ordinare l'espulsione» e avrebbe dovuto anche aggiungere «quando risulta persona pericolosa». Questo è il problema. Se invece si dice «il giudice ordina l'espulsione» sembra che ci sia, invece, una pericolosità presunta.

che solleverà delle eccezioni di costituzionalità e voi direte: ebbene, noi avevamo la volontà di fare questa norma; purtroppo abbiamo trovato degli avvocati che hanno sollevato delle eccezioni di costituzionalità e dei giudici - comunisti, naturalmente - che l'hanno accolta. In effetti, siccome questa norma non riguarda solamente gli stranieri, ma anche i cittadini della Comunità europea appartenenti ad altri Paesi, è in contrasto con l'articolo 27 della direttiva europea 2004/38/CE che dice espressamente che questa pericolosità non può essere desunta esclusivamente da da una condanna penale, così come avete scritto nell'articolo; dice anche, nei successivi articoli 28 e 29,

ad assumere un atteggiamento più rispettoso nei confronti del collega che sta illustrando i suoi emendamenti. Stiamo discutendo di un provvedimento estremamente delicato ed importante.

che introduce una circostanza aggravante comune e come tale applicabile a qualsiasi reato, relativa al fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Essa riguarda quindi un mero *status* soggettivo della persona, privo peraltro di un autonomo disvalore penale, se non di qualsiasi disvalore. Questa mattina, signor Presidente, lei ha commemorato le 140 vittime; se queste 140 persone fossero arrivate in Italia, avrebbero avuto il disvalore

che sono un'altra piaga, perché i clandestini che muoiono sul lavoro si trovano in una situazione di irregolarità. Quindi, basta questa situazione personale per l'aggravante. Questa circostanza, nella misura in cui cui riconduce l'aggravamento della pena prevista per il reato unicamente alla nazionalità in assenza di alcun collegamento con la condotta, con l'elemento psichico, con il disvalore penale, con il bene giuridico e quant'altro, non è compatibile con il principio di ragionevolezza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione,

alla disciplina dell'immigrazione, perché è caratterizzata da carenza di offensività e di assenza di proporzione tra pene e reati. In tale sentenza, la Corte ha invitato il legislatore ad astenersi dall'introdurre dall'introdurre norme che prescindano «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili» o che prevedano sanzioni «tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di eguaglianza e proporzionalità». La relazione tra la nazionalità del soggetto attivo ed aggravio sanzionatorio pare poi nettamente in contrasto con il principio di eguaglianza «senza distinzioni», tra l'altro, di «condizioni personali», sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e con il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È evidente, inoltre, che il riferimento fatto alla norma in esame al «soggetto» e non allo «straniero» la rende applicabile anche al cittadino dell'Unione europea che soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato. L'aggravante, quindi, nei confronti dei cittadini comunitari - nella misura in cui, sia pur indirettamente, ostacola il pieno esercizio del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione europea - appare incompatibile con la direttiva 2004/38/CE, che, com'è noto, ammette limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari solo per ragioni tassative, sufficientemente gravi e in virtù di misure proporzionate e non discriminatorie. I profili di dubbia legittimità della norma sinora illustrati sembrano confermati dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da taluni giudici, chiamati ad applicare la disposizione di cui all'articolo 1,

Questa modifica s'impone anche perché, con i progetti di legge che sono in fase di esame sulla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, verrà esteso l'ambito d'indagine alle mafie straniere. Come sapete, la Direzione investigativa antimafia, nelle sue relazioni semestrali, ci informa sul grado di pericolosità di tali associazioni criminali straniere, cosiddette allogene (in particolare quelle russa, albanese, cinese, rumena, nigeriana, sudamericana, nordafricana e bulgara).

l'emendamento 1.5, da noi proposto, si riferisce all'introduzione di specifiche ipotesi di reato per quei fenomeni criminali che, nel corso degli ultimi anni, hanno destato maggior preoccupazione. Nell'ambito di un decreto che affronta questa tematica, ossia il grave allarme sociale determinato da alcuni fenomeni, ci pareva assolutamente ingiustificato il mancato esame di altre ipotesi criminali che hanno appesantito il nostro Paese e che determinano In modo particolare avevamo richiamato l'attenzione sul fatto che esiste un enorme numero di reati che vengono commessi nell'ambito di quella che dovrebbe invece essere una naturale difesa dell'individuo, ossia la famiglia. Proprio nell'ambito della famiglia si verifica un gran numero di reati.

persone che vivono nel nostro Paese in condizione di irregolarità. Mi riferisco allo sfruttamento dei minori nell'accattonaggio; dietro ai minori ci sono gli adulti.

spesso proprio da parte del genitore, era una condizione che ritenevamo importante inserire in un decreto che affrontava determinate tematiche.

Un'altra ipotesi delittuosa rispetto alla quale il nostro Paese è in notevolissimo ritardo l'inserimento della disciplina degli atti persecutori, cioè di quei comportamenti che presi singolarmente non superano la soglia dell'illiceità e della punibilità ma che visti nel loro complesso costituiscono un grave attentato alla libertà morale e spesso fisica della persona. tratta di comportamenti idonei a distruggere l'esistenza quotidiana di una persona, rispetto ai quali oggi il nostro sistema non è in grado di intervenire perché sono condotte che sfuggono all'incasellamento in una ipotesi specifica di reato. Allora l'inserimento di queste condotte per consentire

Purtroppo il ritardo con cui affrontiamo tale problema ci ha portato in passato a dire che se avessimo fatto ciò avremmo qualche morto in meno sulla coscienza. Pensavamo di poter dire al Paese e al Parlamento che quantomeno noi abbiamo fatto il possibile per evitare altre vittime come quella che pochi mesi fa si è registrata a Genova a seguito proprio di questi comportamenti che non hanno consentito interventi. Invece si è detto che così facendo appesantivamo il decreto; noi non vorremmo appesantire la nostra coscienza con la distrazione e con un ritardo di anni. Come non rispondere ora, in questo momento, attraverso questo reato condiviso? Nella scorsa legislatura l'esame parlamentare nelle Commissioni aveva

non è stato possibile farlo nelle Commissioni riunite, riproponiamo l'emendamento alla sensibilità di questa Aula ritenendo che tali ipotesi di reato possano e debbano trovare

Mi riferisco in particolare all'emendamento 1.23, che si occupa dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Orbene, la violenza domestica è una delle principali cause di morte per le donne in tutto il mondo. In Italia ogni tre giorni, forse anche meno, muore una donna uccisa per mano del proprio *partner,* attuale o *ex*. Se avvenisse tra Paesi - scrivono gli uomini in una dichiarazione «Lega del fiocco bianco» - la chiameremmo guerra, se si trattasse di una malattia la definiremmo epidemica, di una perdita di petrolio un disastro. Poiché accade alle donne è solo una faccenda di tutti i giorni. Vorrei rappresentare, tra l'altro, che

ha introdotto la criminalità nei confronti delle donne come una delle principali preoccupazioni che destano, da una parte, allarme sociale e, dall'altra, richiesta di sicurezza da parte delle donne e dei cittadini in generale.

Il dato sconfortante è che si muore più per violenza domestica che per mafia. Questi dati sono stati ripresi anche recentemente dall'indagine Eures-ANSA e sono assolutamente in linea con quelli che l'ISTAT ha fornito in una ricerca multiscopo sulla violenza e sulla sicurezza delle donne, che è stata commissionata dal Ministero dell'interno con i fondi del PON sicurezza e dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Sulla base della denunzia dell'ISTAT, sono stimate in 6.743.000 le donne da 16 a 70 anni vittime di violenza fisico-sessuale nel corso della vita.

Voglio ricordare, rispetto a quanto ha già riferito il senatore Li Gotti, che proprio recentemente, nel maggio di quest'anno, conseguenza di un'ulteriore ipotesi di *stalking*. A Torino, un uomo, una guardia giurata, ha ucciso l'ex moglie adoperando la pistola che gli era stata prima sequestrata, a seguito della denunzia della moglie, e poi restituita. Le violenze, per quanto riguarda l'anno 2007, da una prima stima, ammontano a circa 126 omicidi, ma si tratta soltanto di una stima giornalistica. omicidi e due tentati omicidi (mi riferisco al periodo che va dal 18 maggio ad oggi). Questi dati sono assolutamente allarmanti e richiedono quindi che si intervenga nel maltrattamento contro familiari e conviventi aggravando le pene previste sia per la fattispecie di base, sia per la prima delle ipotesi aggravate, in particolare portando la pena fino a sei anni e consentendo che si possano effettuare intercettazioni ambientali, affinché le donne non siano lasciate sole a testimoniare e condannate, se ritrattano, anche per calunnia. Abbiamo previsto inoltre di inserire l'ipotesi di atti persecutori come lo *stalking*. Si tratta di una gravissima lacuna nel nostro ordinamento. È una fattispecie che prevede un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari. Ciò potrà in molti casi contribuire ad evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso parla la cronaca. Abbiamo previsto inoltre, per quanto riguarda gli stupri, che costituiscono anch'essi una fetta importantissima della violenza contro le donne, (faccio presente che il Ministero dell'interno dedica ben 40 pagine del rapporto alla violenza contro le donne,

anche alle ipotesi in cui l'autore sia responsabile di gravissimi reati, quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.

Inoltre, abbiamo previsto la specifica aggravante per la commissione del reato di violenza sessuale ai danni di donne in stato di gravidanza: è allarmante il fenomeno che si sta verificando dell'abuso nei confronti di donne incinte che poi abortiscono. È una richiesta che è stata individuata anche nell'ambito del fenomeno della tratta degli esseri umani, poiché la prostituzione minorile viene sfruttata anche sotto questo aspetto. 1 del decreto-legge, abbiamo chiesto che sia comminato l'ergastolo nel caso che l'omicidio avvenga in occasione della commissione dei seguente reati: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,

sul triste episodio che ha riguardato il tenente dei carabinieri Marco Pittoni, ucciso pur disarmato. L'emendamento 1.729, composto da sole tre righe e che si illustra da sé, in realtà ha un profondo significato: l'Italia si comporta nei confronti delle forze dell'ordine, talvolta per una sua piccola parte, in modo certamente diverso da come si comportano Francia, Germania, Inghilterra. Paese non c'è la certezza della pena e tante volte le pene, pur essendoci, in qualche modo non sono scontate in virtù di tutta una serie di provvedimenti e di riferimenti normativi a leggi fin troppo permissive.

- come è accaduto la settimana scorsa quando, lo ripeto, un agente disarmato è stato barbaramente ucciso da chi è stato definito balordo sui giornali ma è delinquente già condannato, figlio di un capo camorra -

non solo di animo ma di razionalità nel comprendere che le forze dell'ordine vanno meglio tutelate. Pertanto, la proposta di aggiungere all'articolo 576 del codice penale la previsione dell'ergastolo per chi uccide un componente delle forze dell'ordine non credo dovrebbe trovare

riferimento all'introduzione dell'aggravante della condizione di irregolarità dello straniero nel nostro territorio. Noi riteniamo che sia giusto che sia giusto l'inasprimento della pena nei confronti di chi si trova irregolarmente nel nostro Paese, ma si deve trattare di uno stato di irregolarità qualificata.

più frequenti è quella della scadenza del permesso di soggiorno o della scadenza del contratto di lavoro del cittadino extracomunitario.

dai ritardi con cui l'amministrazione dello Stato procede all'esame delle domande per il rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche dalla rigidità del sistema del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro extracomunitario. Non qualificare lo stato di irregolarità nel momento in cui si introduce questa aggravante significa sostanzialmente introdurre un aggravamento indiscriminato

che noi proponiamo con l'emendamento 1.3, in base al quale il meccanismo dell'aggravante scatta solo nel caso in cui il soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale si sia sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. perché ciò che costituisce il presupposto è la condotta e la condotta in questo caso è riconducibile alla circostanza che il soggetto si sia sottratto ad un ordine dell'autorità. Si tratta peraltro di una disposizione di buonsenso che si inserisce in maniera molto più coerente nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto dal nostro codice penale e che, per altro verso,

valutabile ai sensi dell'articolo 62-*bis* del codice penale quale circostanza attenuante generica. La circostanza che un soggetto che commette un reato

c'è una pratica diffusa, generalizzata e sostanzialmente non motivata, relativa alla diminuzione dell'apparato sanzionatorio penale fissato dal legislatore, con riguardo ovviamente alla giurisprudenza, atteso che è notorio che le cosiddette attenuanti generiche ormai rappresentano una diminuzione fissa della pena, senza sostanziale valutazione di elementi concreti a favore del condannato. L'idea che il soggetto che commette un reato, indipendentemente dalla gravità del reato, indipendentemente dalla modalità della condotta, indipendentemente dal contesto in cui questa condotta opera, solo per essere incensurato ottenga uno sconto di pena

da parte delle unità militari locali e italiane, ha ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, tant'è vero che da quando è entrato in vigore questo patto bilaterale dall'Albania non c'è stata alcuna nave o gommone che abbia raggiunto le coste italiane.

sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente se non addirittura al loro interno. Pertanto la Lega invita il Governo ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale dai clandestini, nonché ad intensificare iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente dei flussi diretti verso le coste del nostro Paese. Solo così si eviteranno grandi e nuove tragedie come quella dei 150 clandestini morti nel Mediterraneo. Aiutiamoli a casa loro, è la soluzione migliore; prendiamone atto tutti.

ho il dovere di far sentire la voce della mia isola e, al contempo, di lanciare un messaggio ai colleghi di sinistra che in questo mese ho ascoltato abbondantemente al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Basta con la sconsiderata politica immigratoria di questi ultimi anni! Basta con questo falso e dannoso buonismo, non se ne può più! Soprattutto noi lampedusani non ne possiamo più!

tranne qualche collega della Lega che in questi anni è stato solidale con i problemi di Lampedusa e non solo riguardo al fenomeno dei clandestini, lo si deve sapere. del giorno G1.101 - circa 7.000 clandestini sono stati soccorsi con la nostra legge sbagliata. Infatti, cari colleghi, a Lampedusa non ci sono mai stati veri sbarchi

Non vi permettiamo di criticare il lavoro che stiamo svolgendo e le misure che intendiamo applicare, perché non solo salveremo la vita di questi poveri disgraziati, ma soprattutto salveremo la nostra vita. Credetemi, cari colleghi, questa gente va aiutata nella propria terra. Cari colleghi di sinistra, vorrei aggiungere un'altra

Per otto mesi in qualità di amministratore locale vi ho chiesto di costruire le scuole a Lampedusa e avete fatto orecchie da mercante. Per un anno i miei figli e quelli dei miei concittadini sono andati a scuola nel plesso della Chiesa: vergognatevi, perché ve l'ho ripetuto per otto mesi!

perché hanno bisogno di dialisi. È da vent'anni che sono costretti a vivere lontano da Lampedusa. Vergognatevi ancora!

Sapete che esiste un'isola che si chiama Linosa? Qualcuno mi ha detto, ma cos'è qualcosa da mangiare? No, è un'isola in cui vivono 500 persone,

Signori rappresentanti del Governo, sto esternando questa mia rabbia,

Una cosa è certa, questo massacro deve finire. Cari colleghi, se non siamo in grado di bloccare tale fenomeno Lampedusa diventerà ancor di più il ventre molle dell'Europa.

qualcosa di sensato. Abbiamo cercato nella discussione della Commissione più volte di sottolineare che è molto importante in termini di immigrazione intervenire non soltanto con norme più severe (se esso siano poi efficaci è tutto da dimostrare), quanto anche sul terreno della prevenzione, soprattutto dal punto di vista degli accordi internazionali. L'ordine del giorno G1.102 chiede al Governo di muoversi in tale direzione stipulando accordi internazionali con i Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso e anche con gli altri, per far sì che, per esempio, le pene possano essere scontate nel Paese di origine e che sugli ingressi vi siano

senza peraltro ricorrere né all'aggravante, né appunto all'introduzione di fattispecie di tipo penale. Questo ci dimostra che, oltre a norme più severe, bisogna fare norme efficaci e lavorare molto su altri versanti per fare sì che non si approvino norme manifesto ma producano risultati concreti. perché, dopo l'intervento sensato della senatrice Incostante, vediamo un'altra insensatezza, che però è una cronaca costantemente riportata e attuale. Succede che nella celebrazione dei matrimoni civili si verificano spesso situazioni anomale che hanno fatto emergere come alcuni di questi sposi non possedevano i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale; si è trattato spesso di matrimoni con giovani donne neocomunitarie, rumene in modo particolare, o con giovani donne italiane, convinte al matrimonio con promesse di denaro, o peggio, di violenza. L'ordine del giorno G1.103, nella sua semplicità vuole solo invitare il Governo ad emanare immediatamente, attraverso le prefetture, le prefetture, una circolare agli uffici dello stato civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del codice civile, nel senso che lo straniero che voglia

questa celebrazione, ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri. Oggi per potersi sposare in Comune

Presidente, mi permetterà un intervento sull'ordine dei lavori. Sarò abbastanza breve, ma credo che il tenore delle comunicazioni che penso di avere il dovere di trasmettere a quest'Aula sia importante ed integri la discussione di questa mattina, che si è incentrata, con qualche tono polemico, sulla lettera del Presidente del Consiglio dei ministri indirizzata a questa Presidenza.

che a proposito dei toni inquieti usati dal Presidente del Consiglio relativamente all'azione della magistratura milanese ai suoi danni, la corte d'appello di Hong Kong ha confermato una decisione dall'Alta corte di emettere una rogatoria per sentire a Milano in qualità di testimoni i pubblici ministeri Fabio De Pasquale, Sergio Spadaro e due loro consulenti in merito all'attività svolta a Hong Kong nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri relativi ai diritti TV di Mediaset. In questa inchiesta sono coinvolti un mediatore, ed il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che viene accusato di essere stato il socio occulto nella compravendita di diritti televisivi e cinematografici. la corte di appello di Hong Kong ha chiarito che sarebbe essenziale che i quattro componenti del *team* della pubblica accusa italiana, andati a Hong Kong contro ogni tipo di giurisdizione internazionale) a svolgere perquisizioni e perfino interrogatori, fossero sottoposti a controesame sotto giuramento, circa la legittimità dell'attività svolta a Hong Kong presso uffici ed abitazioni di società e dirigenti sottoposti a perquisizione con sequestro di vari documenti cartacei ed informatici. Secondo le notizie che giungono da Hong Kong (mi permetto

abbia deciso sul punto immediatamente, in udienza, anziché riservarsi, come avviene nella quasi totalità dei casi consimili. Le inquietudini del presidente del presidente del Consiglio Berlusconi, dunque, sarebbero clamorosamente confermate anche da questa notizia, che io chiederei alla Presidenza ed al Ministro della giustizia di voler approfondire, perché siamo di fronte ad elementi che lasciano immaginare una vera e propria persecuzione nei confronti di un'alta carica dello Stato. La stessa cosa è avvenuta in un altro Paese del mondo: del mondo: la corte distrettuale della California ha annullato un sequestro effettuato a Los Angeles, ordinando la restituzione di tutto il materiale e vietando la trasmissione delle carte ai pubblici ministeri di Milano. Anche un'analoga rogatoria avviata in Irlanda sarebbe stata infruttuosa e nessun documento sarebbe stato consegnato ai pubblici ministeri italiani. Quando il presidente Berlusconi parla di persecuzione ai suoi danni,

abbiamo presentato questo ordine del giorno insieme ai colleghi della delegazione radicale, senatori Bonino e Perduca, per anticipare un dibattito che, per certi versi, si era già aperto con

legge già arrivato al Senato. Allora, visto che comunque questo decreto-legge parla di sicurezza, di ordine pubblico e del diritto penale, prevedendo misure per contrastare e prevenire la criminalità

i nostri cittadini italiani, quelli buoni e con passaporto italiano, vanno a comprare del sesso a pagamento. Se questa è la situazione, forse è il caso di intervenire pensando di togliere del denaro a questa criminalità organizzata, come avvenuto in gran parte dei Paesi dell'Unione europea, dove è stato fatto un discrimine cosa è legale e cosa non lo è. Non è legale sfruttare una donna e ridurla in schiavitù per strada; è legale che una donna o un uomo maggiorenni possano decidere di fornire prestazioni di attività sessuali a persone, ovviamente maggiorenni, e purché tutto questo avvenga tra persone consenzienti. È inutile che mi guardi così, senatore Berselli! Lei pensa di intervenire con una bacchetta magica e che immediatamente tutti gli uomini italiani non vadano più a prostitute lei ha deciso che prostituirsi per strada da parte di una donna immigrata clandestina è un reato, un aggravante e così la può espellere; io invece non credo che con la bacchetta magica dell'emendamento si risolvano grossi problemi, fenomeni sociali esistenti non solo in Italia ma in tutto il mondo. me, è bene separare la prostituzione volontaria da quella coatta e far sì che l'apparato repressivo

come un lavoro, esistono ancora molte situazioni in Europa dove le *sex workers* sono discriminate e senza diritti. La prostituzione è ormai un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzarne i diritti. Onorevoli colleghi, credo che governare i fenomeni sociali sia davvero più efficace che proibirli. Un fenomeno sociale, appunto, si governa, si gestisce e non si fa scomparire a colpi di proibizioni. diverso se si possedesse la bacchetta magica, ma a meno che il Presidente del Consiglio non si trasformi nella vignetta di Giannelli e con il cappello magico e con la bacchetta faccia davvero scomparire le prostitute dalle strade italiane, credo che, come nel caso dell'immigrazione, non è certo con la bacchetta magica che si faranno scomparire i morti e i clandestini che continuano ad arrivare sulle coste italiane, ma

sono privi di portata modificativa.

del complesso denominato «pacchetto sicurezza» vi sono disposizioni che disciplinano il contrasto e la prevenzione dei cosiddetti matrimoni di comodo. Il Governo si rende conto che non è la stessa materia

che ci ha aiutato moltissimo nel nostro Paese ad individuare le caratteristiche tipiche dell'organizzazione mafiosa e a colpirla in quanto tale.

sostenne la necessità che nel nostro ordinamento fosse inserita una norma con tali caratteristiche. Il Parlamento intervenne successivamente, il 13 settembre, e finalmente

Allora prevalse l'antimafia del giorno dopo; non riuscimmo ad esprimere l'antimafia del giorno prima. Ora con questa disposizione si prova a fare un piccolo passo in avanti. È stato necessario provare

ad una richiesta che è stata spesso avanzata nelle varie Commissioni parlamentari antimafia dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, dagli operatori

quando ho espresso il mio disappunto per il cambiamento di rotta e di metodo da parte dei Presidenti delle Commissioni, con cui avevamo lavorato lealmente e proficuamente in questo inizio

ma utilizzando la testa, evitando le impostazioni demagogiche, evitando le norme manifesto, pensando a colpire i comportamenti e non già lo *status* personale dei soggetti interessati dalle norme penali. Quando dico "punire i comportamenti" alludo al fatto che queste disposizioni inaspriscono significativamente le norme in materia di false dichiarazioni. Naturalmente pensavamo in particolare alle false dichiarazioni dei soggetti clandestinamente presenti nel nostro territorio, che si sottraggono all'attività di controllo sbarazzandosi dei documenti, fornendo false generalità e, a volte, addirittura praticando praticando automutilazioni sui polpastrelli in modo da non poter essere identificati con le impronte digitali. Norme severe, norme rigorose, norme costituzionalmente compatibili, norme che colpiscono comportamenti, non lo *status* personale. Devo aggiungere qualcosa nel concludere la mia dichiarazione di voto su questo punto. Ipotizzo un'associazione criminale che si occupi di produrre e fornire a clandestini documenti falsi. Ipotizzo le indagini su questa associazione criminale (ne esistono, lo assicuro). Ipotizzo l'impossibilità, se e quando le nuove norme in materia di intercettazioni dovessero entrare in vigore, di svolgere indagini sulle associazioni criminali che favoriscono, con falsi documenti, la permanenza dei clandestini nel nostro territorio nazionale. Ricordatelo, signori della Lega!

norme molto severe per alcuni reati che suscitano particolare allarme sociale. Rispetto ad alcuni di essi si tratta di vere e proprie emergenze.

penso soltanto al caso dell'accattonaggio, quello che vediamo tra l'altro ogni giorno nelle strade di qualunque città italiana - e per i maltrattamenti a danno di familiari e conviventi. I relatori hanno dichiarato, ad onor del vero, di apprezzare il senso di questi emendamenti, però hanno ritenuto che la materia non fosse strettamente inerente al decreto-legge che stiamo convertendo. Ora, alla luce di quello che sta succedendo, mi permetto di chiedere ai relatori, ma anche ai colleghi della maggioranza, di voler considerare con più attenzione questo aspetto. Se ritenete in qualche misura inerente al tema del decreto-legge la materia di cui stiamo trattando e di cui si legge sui giornali,

in esame l'adescamento dei minori o, ancora peggio, i maltrattamenti per avvengono in famiglia. Pertanto, associandomi alla richiesta del senatore Bianco, chiediamo al Governo

si affermò che allargava l'oggetto del provvedimento. Oggi, dopo che il Governo e i relatori hanno presentato alcuni emendamenti nuovi, ad esempio quello sulla riorganizzazione dei processi e quello sull'impiego dell'Esercito, è ovvio che, essendosi ampliata la materia,

Presidente, credo che sia superfluo richiamare quello che il Governo, uniformandosi anche agli interventi dei relatori, ha già detto in Commissione. Vorrei solo ricordare che il provvedimento sullo *stalking*, di cui vi è traccia nell'emendamento 1.23, su cui prima si è soffermata la senatrice Della Monica, è già incardinato presso la Commissione giustizia della Camera

con l'ordine dei lavori parlamentari rispettare quanto è già stato avviato nelle sedi opportune e lo stesso vale per l'accattonaggio che trova sede nel disegno di legge.

urgenti; sono tutti settori che riguardano la sicurezza pubblica sui quali bisogna intervenire adesso e non c'è nessun motivo per rinviare decisioni su questo argomento.

anch'esse necessarie e urgentissime, talmente urgenti da essere state fatte rientrare in un decreto che ha finanziato le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Norme veramente urgenti che hanno poi aperto la strada due anni fa a tutta un'altra serie di urgenze poi incluse in questo decreto sicurezza.

l'argomento è importante vorrei ricordare soltanto che la legge, giustamente, non è stata modificata nei due anni precedenti perché con il senatore Marino e altri senatori e deputati avevamo convenuto

per chi guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, e quindi in grado di nuocere a se stesso ed agli altri, sono previste sanzioni, quali la confisca, che penso possano essere ampiamente condivise. Solo per gli spacciatori, ricordo, c'è la sanzione penale: ma lo dico perché i giovani che vanno in Grecia, negli Stati Uniti o in Francia possono trovarsi in galera anche per uno spinello. In Italia ciò non avviene: abbiamo una legge civilissima che distingue i consumatori, vittime, e gli spacciatori, che invece vanno perseguiti. Naturalmente tutto è perfettibile, ma questa versione di questa fantomatica legge che criminalizza i giovani non esiste. Ricordo che a livello di Nazioni Unite le droghe leggere e quelle pesanti sono nella stessa tabella e che tutti i rapporti internazionali, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, ricordano che nella *cannabis* i princìpi attivi sono aumentati ad un livello tale da essere gravemente nocivi della salute soprattutto dei giovani. Non ci sono droghe leggere o pesanti: ci sono droghe e basta, che fanno male e vanno in qualche modo

che è alla guida abbia assunto tali sostanze e sia sotto il loro effetto non è poi così semplice, perché se da un lato abbiamo l'etilometro

sia avvenuto perché in quel momento non ero in grado di guidare o non ero in grado di avere una piena coscienza di me, del mezzo e di quello che stavo facendo. Quindi, sottoporrei davvero all'attenzione dell'Aula, e in caso anche del Governo, l'opportunità una strumentazione che sia utile a dimostrare che il soggetto effettivamente era sotto l'effetto di stupefacenti, cosa che non è così facile con i test che esistono oggi in circolazione, tenere conto delle sostanze: per la cocaina vale un discorso, per la *cannabis* un altro, esiste tutta una serie di gradazioni, e in qualche modo bisognerà prevedere come intervenire.

fatto tutto nell'arco di un batter di ciglio e non si è visto niente. Qui c'è un resoconto stenografico, non di immagini, ma io non ho visto nessuno che alzasse la mano. È stato detto «favorevoli, Siccome si tratta di provvedimenti necessari ed urgenti secondo il Popolo della Libertà, bisognerebbe applicare sistematicamente il oltre che dell'urgenza, di avere un dibattito relativo a tutto ciò che cerca di migliorare queste pessime norme, ma se non altro, poi, si dovrebbe farle votare in maniera tale che tutti possano esprimere il proprio parere. parere. Spero che si possa trovare qualche anima pia in quest'Aula che abbia fatto delle foto o abbia ripreso delle immagini nel momento in cui è stato posto ai voti il mio emendamento. Il senatore Giovanardi nella sua replica ha detto cose cose evidenti, perché da 40 anni sono evidenti i fallimenti delle politiche proibizioniste portate avanti dalle tre Convenzioni delle Nazione Unite in materia di sostanze stupefacenti. Non esiste un documento scientifico prodotto dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione mondiale della sanità, o dall'Agenzia per le droghe e il crimine di Vienna, in cui scientificamente si riesca a fare la distinzione fra le piante

e il prodotto raffinato che effettivamente può avere, se assunto in determinate quantità (e non da tutti allo stesso modo ma individualmente), degli effetti tossici. L'esempio fatto dal senatore Giovanardi, relativamente alla *cannabis*, si alla *cannabis*, si rifaceva ad articoli di stampa dell'«Independent», un giornale che dieci anni fa aveva svolto una campagna a favore della legalizzazione della canapa indiana e dei suoi derivati

si sono arricchite! Sono 40 anni di valore aggiunto a delle sostanze che di per sé non ne avrebbero; 40 anni che hanno creato un clima criminogeno che voi, portando avanti la legge che reca il nome del ministro Giovanardi e la legge Bossi-Fini, volete in qualche modo raggruppare per regalarci cinque anni di tolleranza zero

Presidente, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge di conversione del decreto-legge è arrivato in Commissione affari costituzionali ed ha superato il primo vaglio, quello relativo alla sussistenza dei presupposti, abbiamo immediatamente segnalato alla maggioranza e al Governo il nostro orientamento sarebbe stato favorevole alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti perché consideriamo assolutamente urgente che si intervenga con provvedimenti che diano maggiore sicurezza ai cittadini: questa è certamente una delle domande di maggiore forza che viene sottoposta dall'opinione pubblica all'attenzione delle forze politiche. Naturalmente, abbiamo ricordato che molte di quelle norme erano contenute nel decreto-legge che il ministro Amato aveva predisposto e che non fu possibile, purtroppo, approvare nella precedente legislatura, ma la questione in oggetto dell'aggravante ritenemmo fosse una delle questioni più delicate ed importanti. L'emendamento che stiamo considerando è un emendamento non soppressivo, come ha detto assai opportunamente il collega D'Ambrosio, ma che risponde ad una logica che è di sistema. Si tratta cioè di colpire con durezza quegli immigrati clandestini che sbagliano, che si trovano nel territorio nazionale e che non rispettano le leggi. E nell'ambito del sistema delle aggravanti ne viene prevista una così come viene prevista per coloro i quali sono in uno stato di latitanza - specifica per coloro i quali, espulsi dal territorio nazionale, continuino a stare in Italia in modo illegittimo: andiamo a colpire con fermezza nell'ambito, però, di una norma che ha una portata di carattere generale. In quell'occasione, con un atteggiamento costruttivo da parte della Commissione affari costituzionali e della sua maggioranza, fu dichiarato che la nostra richiesta era assai ben fondata. Ad un certo punto abbiamo percepito che nella maggioranza o nel Governo era immotivatamente cambiata opinione su questo punto. Vorremmo invitare i colleghi della maggioranza a considerare con la dovuta attenzione questo emendamento perché sicuramente colpisce con fermezza coloro i quali - ripeto si trovano in Italia espulsi e non dovrebbero starci, ma si muove nell'ambito di un quadro di sistema. Quindi noi chiediamo con forza ai colleghi di valutare con attenzione una posizione che certamente è assai rigorosa. [LI

si specifica che le circostanze inerenti la persona del colpevole sono quelle attinenti alla recidiva e alla imputabilità e non ad altre. ad altre. Fermo restando l'articolo 70 del codice penale, ultimo comma, l'introdurre un'aggravante inerente la persona del colpevole con la lettera *f*) crea un profilo di palese assurdità normativa e sistematica del nostro codice, oltre a porsi in contrasto con pronunzie già intervenute da parte della Corte costituzionale la quale, anche con la recente sentenza n. 192 del 2007, ha affermato come l'assenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmente irrilevante ai fini del disvalore dell'azione, che va desunta dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere, secondo i criteri di cui all'articolo 133. Le condizioni di reità, così assimilandosi la condizione di irregolarità - questo è il processo logico seguito dal Governo - sono già previste dall'articolo 61 del codice penale. Sono previste due specifiche aggravanti al numero 2) e al numero 6). Al numero 2) si prevede la condizione di precedente reità, pur richiedendosi la necessità del nesso teleologico tra il nuovo fatto commesso e la condizione di reità.

introduce l'aggravante collegata non tanto alla reità quanto

In sostanza, la condizione di reità di per sé non è aggravatrice della condotta del successivo reato ma lo è la misura cautelare emessa per il precedente reato.

tant'è vero che il reato e l'aggravante sussistono anche qualora per il fatto per il quale era stata emessa la misura cautelare intervenga l'assoluzione: ciò ciò che si sanziona, cioè, è il comportamento di ribellione ad un ordine dato dall'autorità. E allora, se questi sono i presupposti che considerano le condizioni di reità, come può inserirsi

È palese l'incostituzionalità. Avevamo offerto una soluzione ragionevole, nel senso di non perseguire assolutamente quella strada. Colgo una volontà della maggioranza e del Governo di imbattersi nei profili di costituzionalità: l'ha fatto con le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1; lo rifà con la lettera *f)* dell'articolo 1. volersi scontrare con pronunzie di costituzionalità che sono già state emesse, quando è possibile trovare la soluzione più ragionevole, che protegga, tuteli e renda efficace questa norma, che condividiamo, ma che vogliamo fatta bene? Questo è lo spirito con cui ci siamo opposti e per questo motivo insistiamo perché il nostro emendamento venga giuridicamente soppesato e non emotivamente votato. Stiamo parlando di diritti e di diritto: cerchiamo di ragionare in termini di legge e non attraverso l'emozione

secondo è che il capo della Polizia, quand'è venuto in audizione nelle Commissioni, ci ha detto che il 70 per cento degli immigrati irregolari nel nostro Paese

clandestinamente con gli sbarchi e quant'altro, mentre abbiamo sempre questa visione dell'immigrazione clandestina con riferimento agli sbarchi. Ora, ci troviamo di fronte alla necessità di mettere anche la magistratura nelle condizioni di intervenire e applicare l'aggravante.

ulteriore. Credo che invece sia più opportuno, più efficace e più produttivo, anche ai fini di coloro i quali propongono l'introduzione dell'aggravante (parlo dei colleghi della maggioranza), qualificarla dicendo che, poiché il soggetto che si trova in condizione di irregolarità irregolarità deve avere un accertamento giudiziale o dell'autorità di pubblica sicurezza, e quindi l'ordine di allontanamento, di espulsione e quant'altro, la sottrazione all'ordine diventa condotta, comportamento che determina l'applicazione dell'aggravante. Tutto questo risparmia tempo alla magistratura, rende più efficace l'applicazione dell'aggravante e su questo aspetto ci ritroviamo tutti quanti. Signor Presidente, sinceramente non riesco a capire perché dobbiamo riferirci a pregiudizi pregiudizi di carattere ideologico anche su questioni di merito assolutamente condivise.

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.700, 8.0.700, 9.702, 12.0.705. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.5, 4.0.100, 5.0.4 e 12.0.702. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 5.0.900, 12.0.300, 12.0.400,

Le innovazioni legislative, invece, vale a dire le modificazioni della legislazione vigente, se danno luogo ad oneri devono, in forza dell'articolo 81 della Costituzione, recare esse stesse le risorse a copertura degli oneri che hanno determinato. Questo significa che un'innovazione legislativa che determini oneri non si può coprire sul bilancio a legislazione vigente, perché la copertura di un'innovazione legislativa onerosa sul bilancio a legislazione vigente costituisce un'aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione e come tale è considerata anche dalla nostra legge di contabilità. Signor Presidente,

In buona sostanza, cosa accadrà quando questa norma sarà stata approvata? Bisogna che accada, signor Presidente, colleghi - inesorabilmente perché è così sotto il profilo tecnico

vi sia la notifica, naturalmente a carico della finanza pubblica, a tutti i soggetti impegnati in quei processi dell'avvenuta sospensione per un anno:

corso. Signor Presidente, la domanda è molto semplice: la notifica, in un processo penale, è onerosa per la pubblica amministrazione? La risposta ovviamente è sì. L'attività di notifica è onerosa, tant'è che le spese di giustizia previste nel bilancio servono a coprire anche queste attività. Il bilancio Il bilancio a legislazione vigente per i processi in corso, signor Presidente, ha certamente previsto le risorse necessarie per la notifica avvenuta quando i suddetti processi si sono aperti. Ma come è come è possibile che il bilancio a legislazione vigente abbia considerato un'attività di notificazione per la sospensione di un processo che solo oggi, venisse approvata quella norma, interverrebbe a sospendere per un anno il processo stesso? Bisognerebbe quindi procedere alle notifiche, determinando così un onere doppio rispetto a quello sopportato a carico del bilancio dello Stato in occasione dell'apertura dei processi.

mentre l'innovazione legislativa è onerosa, poiché produce la necessità di moltiplicare le attività di notifica non per due, ma per tre.

ci sarà), non presenta una relazione tecnica che motivi il giudizio sull'indifferenza finanziaria della norma? Il merito viene lasciato completamente impregiudicato. Se avessi ragione io, bisognerebbe introdurre una copertura della norma, se avesse ragione la maggioranza della Commissione bilancio, l'emendamento potrebbe essere votato così com'è, perché non si porrebbero problemi di carattere finanziario.

nostro esame è un emendamento del relatore e questo obbligo formalmente non c'è, tuttavia, signor Presidente, lei questa mattina ci ha letto una lettera del Presidente del Consiglio,

mi permetto di dissentire profondamente dall'intervento del collega Morando, come è avvenuto anche nel corso della riunione della Commissione. Commissione. Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni che il collega Morando ha svolto sia in Commissione che in Assemblea, ma né in quel caso, né in questo, a mio avviso, egli ha addotto ragioni convincenti per supportare la sua richiesta. Devo fare una premessa di ordine

Quindi, sul piano procedimentale è chiaro perché manchi la relazione tecnica; infatti, il Ministro dell'economia, confermando l'assunto degli uffici della Commissione, ha ritenuto l'emendamento non essere oneroso.

non è mai definito il numero di notifiche necessarie. Le notifiche in un processo cambiano per le più disparate ragioni. Basti pensare a quelle della modifica di un collegio piuttosto che a quelle di una nullità, di una dimenticanza dell'ufficio o delle necessità di una delle parti, siano esse la parte pubblica, quelle dei difensori o della parte civile. La notifica in ciascun processo non rappresenta un costo singolo; il costo complessivo delle notifiche è quello previsto a legislazione vigente. All'interno di un costo complessivo e di per sé variabile si inserisce una notifica per la sospensione,

che il costo delle notifiche a legislazione vigente sia precisamente identificato. Tale costo è quello relativo a tutte le notifiche necessarie per lo svolgimento del processo nell'ambito del quale - lo ribadisco - si ricorre alle notifiche per le ragioni più disparate e mai preventivamente identificabili. Per questa ragione il costo è quello complessivamente inteso e l'innovazione a legislazione vigente, che è che è certa, non è tale sul piano dell'onere che - ripeto - è previsto a monte (come è necessario nel nostro caso) per tutte le possibili notifiche che si rendono necessarie in un processo.

sui quali la Commissione bilancio, per prassi consolidata, esprime il parere di nulla osta per la loro non onerosità. Per questa ragione la maggioranza della Commissione ha richiesto di votare l'emendamento il quale ha ricevuto poi il parere di nulla osta della Commissione

processo e non fosse compensata dall'onere generale, essa comporterebbe un onere totalmente trascurabile. Questa, però, signor Presidente, è soltanto un'aggiunta di carattere personale perché ho

legittimo e anche argomentato dissenso dei colleghi dell'opposizione, mi sembra possa essere confermata anche in questa sede.

che, volendo fare anche un altro tipo di considerazione, si potrebbe ipotizzare non solo la non onerosità dell'emendamento, ma anche, paradossalmente, la sua virtuosità, in quanto i processi sospesi non darebbero vita a quella che è l'esigenza fisiologica di notifica di atti e di provvedimenti del collegio giudicante nell'*iter* giurisdizionale. Quindi, questa sospensione potrebbe determinare sostanzialmente delle economie. Ma è soltanto una considerazione squisitamente personale.

Presidente, penso che questa proposta abbia un grande valore umano e culturale per l'Aula, per tutti noi

regalare a questo concittadino così valoroso e così rappresentativo un pensiero di profonda commemorazione.